Onorevoli colleghi, il 20 maggio di 10 anni fa, a pochi passi dalla sua abitazione, cadeva assassinato il professor Massimo D'Antona. Quei sei colpi di pistola, nello stroncare la vita di uno tra i più stimati giuslavoristi del nostro Paese, interrompevano duramente l'ormai decennale illusione che, dopo l'assassinio del senatore Ruffilli, la stagione del terrorismo fosse finita per sempre. Anche questa volta, la vittima era prescelta tra le figure più significative di quella cultura riformatrice che - consapevole della necessità di realizzare strumenti di coesione sociale più adeguati al mutamento dei tempi e al diverso contesto europeo ed internazionale operava per avviare una riforma del mercato del lavoro pubblico e privato, e per costruire nuovi modelli di relazioni sindacali. Professore di diritto del lavoro presso le università di Catania e di Napoli, ed infine presso l'università "La Sapienza" di Roma, Massimo d'Antona fu, prima di tutto, giurista di grande spessore. Dalla monografia sulla reintegrazione nel posto di lavoro e dalla riflessione sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fino al saggio inedito sul quarto comma dell'articolo 39 della Costituzione, che fu ritrovato nella sua borsa crivellata dai colpi degli assassini, ogni suo contributo scientifico mostrava, con lucidità di analisi, la direzione da percorrere per superare le criticità e le carenze del nostro modello sociale. Negli ultimi anni prima della morte, quale concreto perseguimento degli obiettivi di riforma resi evidenti dalla lucidità della sua analisi, all'attività accademica si era affiancata una generosa opera di consulenza - svolta sempre a titolo gratuito -verso il Ministero del lavoro e le Commissioni parlamentari competenti. Tra gli estensori del Patto per lo sviluppo e l'occupazione, siglato nel 1993 tra il Governo Amato e le parti sociali, durante il Governo Dini fu consigliere giuridico del ministro dei trasporti Caravale e, successivamente, venne nominato Sottosegretario di Stato presso il medesimo Dicastero. L'impegno per le istituzioni non era vissuto mai, però, come una pratica a sé, separata dall'elaborazione intellettuale, ma come un completamento necessario della ricerca scientifica, nel quale verificare e realizzare i risultati prodotti della riflessione teorica. In quei mesi del 1999 - gli ultimi della sua esistenza - la collaborazione con le istituzioni del professor D'Antona era concentrata sulla realizzazione normativa dello storico processo di privatizzazione del pubblico impiego, di cui egli può essere, a pieno titolo, considerato uno dei padri. Riforma che poté vedere però compiutamente la luce soltanto due anni dopo la sua morte, con l'emanazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Le idee di Massimo D'Antona, come studioso e come uomo di governo, costituiscono, per noi, un lascito ancora attuale. Sulla riforma della pubblica amministrazione, la sua tenace difesa dell'effettività del processo di privatizzazione del pubblico impiego, nel momento in cui se ne definivano i primi contenuti, e la sua attenzione nei confronti della compatibilità fra i risultati della contrattazione collettiva e gli equilibri di finanza pubblica costituiscono ancora un prezioso riferimento. Ciò risulta di particolare interesse quando, come sta avvenendo nella corrente legislatura, si pone mano a numerosi aspetti della riforma del 2001, al fine di completarne e renderne effettivi i risultati: dalla valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, alla rimozione degli ostacoli che ancora ne rendono problematica la mobilità dall'uno all'altro settore dell'amministrazione centrale o dall'uno all'altro livello di governo; dall'introduzione di strumenti di verifica della professionalità e dei risultati amministrativi, alla valorizzazione dei gradi più elevati della dirigenza pubblica. Per quanto riguarda, poi, il tema più generale dell'evoluzione verso un mercato del lavoro e un modello di coesione sociale più efficace e coerente, rimane di grande attualità l'invito pressante, rivolto dal professor D'Antona al sindacato e a tutti gli attori del mercato del lavoro, a dare la massima attenzione, più che alle masse ed alle categorie, al "lavoratore concreto, in carne ed ossa, al suo progetto di lavoro e di vita". Soltanto un simile "umanesimo del lavoro", del quale Massimo D'Antona è stato tra i protagonisti più illustri, può aprire la strada ad una interpretazione più attuale, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione, soprattutto in un contesto in cui la difficile congiuntura economica rischia di provocare il tentativo, da parte di forze minoritarie, di esasperare irresponsabilmente il disagio sociale. Come egli aveva intuito, è necessario che la tutela del lavoro si trasformi, da garanzia rigida della conservazione del "posto", in una tutela più efficace e flessibile assicurata alla persona del lavoratore e alle sue legittime aspettative di impiego. Soffermarsi sulla grande attenzione mostrata da Massimo D'Antona, nei suoi studi e nella sua attività istituzionale, nei confronti delle singole persone e dei loro destini, non può che provocare ulteriore sdegno e commozione, se si confronta questa dedizione umana con la spietatezza dei suoi assassini. Olga D'Antona, in un'intervista rilasciata poche settimane dopo la morte del marito, pronunciò frasi che ancora toccano il cuore, contro quella "banda di assassini deliranti" che, nel vano tentativo di destabilizzare la nostra democrazia, non sanno fare altro che "colpire delle famiglie, creare dolore privato". "A loro" (sono le sue parole) "non interessano le storie personali, essi non danno alcun valore alla felicità di un individuo. A quali masse informi si riferiscono questi assassini? In nome di quale utopia sparano al cuore di un uomo inerme?" Oggi che quegli assassini sono assicurati alla giustizia, il nostro "sforzo costante per coltivare ed onorare la memoria delle loro vittime", secondo le parole pronunciate dal Capo dello Stato in occasione della giornata della memoria, ci impone non soltanto di ricordare, come stiamo facendo quest'oggi, ma di rendere viva la memoria facendo sì che i valori e le idee di Massimo d'Antona siano ancora presenti in tutti gli sforzi compiuti da maggioranza ed opposizione e dalle forze sociali più attente e responsabili - ciascuno nel proprio ruolo - per costruire un mondo del lavoro più moderno e più giusto. Rivolgo perciò, certo d'interpretare la volontà dell'intera Assemblea, alla moglie Olga D'Antona, a sua figlia Valentina e a tutti i lavoratori che hanno perso con lui un vero difensore, un saluto commosso, nel nome della nostra più profonda vicinanza e solidarietà umana. Invito pertanto l'Assemblea ad un minuto di raccoglimento.

colleghi, questa mattina, nel salone a lui dedicato presso la sede storica del Ministero del lavoro di via Flavia, abbiamo voluto rendere onore alla memoria del professor Massimo D'Antona, assegnando un premio a due giovani impegnati nello studio delle dinamiche del mercato del lavoro e delle relazioni industriali nel pubblico impiego. L'iniziativa di questa mattina, realizzata in collaborazione con la "Fondazione Prof. Massimo D'Antona (Onlus)", ci ha consentito di ricordare la sua attività di studioso e il suo ruolo di docente universitario, tra i più autorevoli e profondi della sua generazione, apprezzato e benvoluto anche per questo dai colleghi e dai suoi studenti. Alimentare il metodo di lavoro e mantenere vivi il pensiero e l'elaborazione scientifica di Massimo D'Antona, che ancora oggi è uno degli autori più citati negli studi sugli snodi cruciali del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, è probabilmente il modo migliore per rendergli omaggio e onorarne la memoria. Oggi ricorre il decennale del suo barbaro assassinio. In questa sede non possiamo non ricordarne, accanto alla preziosa attività di insegnamento universitario, la passione civile e il generoso impegno al servizio delle istituzioni democratiche e dello Stato. Marco Biagi - ha pagato un prezzo inaccettabile per il decisivo apporto offerto alla battaglia per la modernizzazione del diritto del lavoro italiano. Ricordo, in particolare, il contributo alla revisione della normativa sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; la regolamentazione della rappresentanza sindacale nel settore pubblico; l'introduzione in Italia del metodo di coordinamento aperto e per obiettivi nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione e dei relativi piani nazionali di azione; infine, la privatizzazione del lavoro pubblico, che rappresenta probabilmente la sua realizzazione più compiuta sul versante della progettazione normativa, come lei, signor Presidente, Nel mio impegno alla guida del Ministero del lavoro per rilanciare il ruolo delle relazioni industriali in una prospettiva cooperativa e meno conflittuale mi ha colpito leggere uno studio, d'inizio anni Novanta, di Massimo D'Antona sulla partecipazione dei lavoratori, che ritengo oggi di grandissima attualità e rilevanza. Già negli anni Ottanta - rilevava D'Antona in quel saggio - si era formata la consapevolezza, in larghi settori sindacali e politici, che il contrattualismo rivendicativo avesse (cito testualmente) "mostrato il tetto delle sue possibilità" e che si dovessero "ormai studiare forme di democrazia industriale capaci di trasformare il contropotere o potere di veto, detenuto dal sindacato in quanto soggetto conflittuale, in un potere positivo di indirizzo e di controllo". Su questo tema siamo oggi impegnati e valuto con estremo favore la circostanza che, proprio in concomitanza con il decennale della tragica scomparsa di Massimo D'Antona, venga definito, in Senato, un percorso legislativo condiviso sul tema della partecipazione dei lavoratori agli utili e all'attività di indirizzo dell'impresa. poche settimane fa Pietro Ichino, durante la commemorazione di Marco Biagi, ciò che caratterizzava l'impegno e l'elaborazione di Massimo D'Antona, così come di Marco Biagi e dei pochi veri riformisti del lavoro, era la convinzione secondo cui i valori protetti dal diritto del lavoro possono essere difesi efficacemente soltanto se lo si aiuta ad evolvere, ad adattarsi al mutare dei tempi, per poter conservare la propria essenziale funzione. Personalmente ho avuto modo di lavorare con Massimo D'Antona solo in occasione del negoziato con le organizzazioni sindacali sul testo dedicato alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, diventato poi decreto legislativo n. 29 del 1993, che ho avuto modo di promuovere allora, come incaricato al Ministero della funzione pubblica. Mi ricordo bene, però, quanto di lui mi diceva Marco Biagi, che ne ammirava l'equilibrio e lo stile nel condurre trattative non facili con le parti sociali. Marco mi parlava di come, nello spazio di poche ore, D'Antona riuscisse a predisporre soluzioni, anche tecnicamente complesse, a problemi insorti improvvisamente e mi parlava anche della grande versatilità che gli consentiva di offrire un parere, di progettare una soluzione su temi anche lontani tra loro: dal mondo del pubblico impiego alle complesse relazioni sindacali del settore dei trasporti, fino al ruolo di ideatore e regista dell'applicazione delle ultime intese concertative. Doti, queste, che ho visto poi in Marco, nella nostra collaborazione al Ministero del lavoro. Uomini semplici e animati da passione e generosità, che sapevano svolgere un ruolo delicatissimo con un senso dello Stato davvero innato, alla ricerca non della mera mediazione contingente quanto del bene comune e dell'interesse pubblico. È anche per questo che lo hanno ucciso. Massimo D'Antona e chi poi lo ha seguito si sono battuti per questi ideali. Spetta a noi continuare in questo impegno nel suo ricordo e nel suo nome. Colleghi, salutiamo il senatore Hubert Haenel, presidente della Commissione affari europei del Senato francese, che si trova a Roma, in visita ufficiale su invito della Commissione politiche dell'Unione europea del Senato. Il presidente Haenel, durante la sua visita, che prevede vari incontri istituzionali, tra cui quello con il Presidente della Repubblica, approfondirà con la 14ª Commissione i temi dell'applicazione del Trattato di Lisbona e del controllo di sussidiarietà "in fase ascendente" dei progetti di atti comunitari. Signor Presidente, colleghi, è per me particolarmente toccante il ricordo di un intellettuale, un insigne giuslavorista, un professore del quale ho seguito le lezioni nei miei anni giovanili. Il professor D'Antona aveva ricevuto un incarico di insegnamento in diritto del lavoro presso l'università di Catania. Erano, quelli, momenti di grande fermento esistenziale per molti giovani della mia generazione; era l'inizio degli anni Ottanta, con il loro portato di rovine, frutto di sogni infranti, che per molti giovani, purtroppo, si sono tramutati nel mostro del terrorismo, che andava sviluppandosi e germinando nel nostro Paese. In Sicilia, poi, rimaneva pesante e concreto un altro mostro: la mafia, col vigore della sua violenza e della sua cultura che tentava di infiltrarsi nei gangli più riposti della società civile, della politica e delle istituzioni. Per molti di noi l'università era un luogo dove cercare un senso alle cose, risposte a tante domande, a dubbi e a inquietudini. Il professor D'Antona appariva come un intellettuale che sapeva intrigare ed umanamente era affascinante, unendo unendo a un rigoroso razionalismo di stampo sabaudo, da parte di madre, una solarità ed umanità del tutto mediterranea, trasmessagli dal nonno paterno, emigrato a Roma dopo il terremoto di Messina del 1908. Catania e la Sicilia per lui erano un personale viaggio di ritorno. Tale è il mio ricordo come allievo, ma anche di tanti altri che lo conobbero e apprezzarono in quegli anni. Era uno di noi che ritornava e che cercava anche di comprendere le grandi contraddizioni storiche ed umane dei siciliani. Ci tengo a sottolineare la sua figura di professore universitario, il suo impegno con i giovani, la sua capacità di trasmettere sapere. Delle tante parole dette su di lui, dei tanti ricordi, credo che non si sia sufficientemente messo in rilievo quella che fu di gran lunga la sua attività prevalente, quella di studioso. Egli intendeva l'università secondo un modello di tipo stanziale, efficiente, tecnologicamente avanzata, aperta all'esperienza comparata, interattiva con gli studenti e molto comunitaria. Era un maestro per vocazione, di quelli che tutti gli studenti ed i giovani che intraprendono la carriera universitaria si augurano di incontrare. Massimo D'Antona possiamo considerarlo un giurista che operava già nella conoscenza e nella coscienza del nuovo secolo. Gli studi sul mercato del lavoro e sul diritto comunitario, sui vari momenti del rapporto di lavoro, sui nuovi rapporti atipici segnarono una delle fasi più importanti della sua attività scientifica. A queste attività di ricerca si affiancò un'intensa partecipazione all'attività legislativa. In questa opera, con la quale cercava di collegare interpretazione della legge e attività contrattuale, cercò di realizzare una figura compiuta di giurista che non si accontenta di interpretare, ma intende sporcarsi le mani, partecipando direttamente al processo legislativo e politico. Il complesso della sua opera e del suo agire, da intellettuale e da studioso, non è caratterizzato dal compromesso. D'Antona non ha mai cercato il consenso delle parti. Le sue scelte da intellettuale sono sempre state precise scelte di campo. Ha sempre proposto interpretazioni della legge che consentivano una più intensa ed effettiva tutela dei lavoratori. Si trattava sempre di interpretazioni sorrette da una rigorosa coerenza di metodo e quindi da una equilibrata consapevolezza degli interessi in campo. Interpretazioni rigorose che alimentando il dibattito hanno contribuito a far progredire la scienza giuslavorista. D'Antona ha sempre attribuito un valore fondamentale al presupposto di un più ordinato processo produttivo, inteso come valore della comunità civile e condizione necessaria per l'effettiva per l'effettiva ed equilibrata realizzazione di tutti i valori costituzionali. La scelta del patto sociale e della concertazione; la scelta del rafforzamento di un sindacato che possa sintetizzare una vera investitura della base con un'adeguata legittimazione della rappresentanza; la scelta di una più effettiva tutela dei diritti costituzionalmente protetti nello sciopero dei servizi pubblici essenziali; la scelta dell'abolizione di uno Stato sociale di tipo risarcitorio e della sua sostituzione con il miglioramento delle possibilità offerte dal mercato del lavoro non sono scelte di compromesso, nemmeno dal punto di vista politico. Con quelle scelte non si propone uno scambio tra gli interessi delle imprese, dei lavoratori occupati e di quelli inoccupati e disoccupati. Si tende semmai a soddisfare l'interesse pubblico con l'ordinato svolgimento del processo produttivo in una più larga prospettiva, con l'esigenza fondamentale di un ordinato svolgimento della vita civile. Merito di Massimo D'Antona è di aver individuato le coerenti motivazioni culturali e i riferimenti di tecnica del diritto che sorreggono tali scelte. È quindi un dovere da parte nostra ricordare oggi chi ha pagato con la vita per il suo impegno civile, come ha voluto sottolineare molto autorevolmente ieri il Capo dello Stato Giorgio Napolitano. È importante saper trasmettere alle giovani generazioni di oggi il ricordo delle tante, troppe vite spezzate dalla cieca e crudele violenza del terrorismo politico. È un obbligo e un dovere da parte nostra riaffermare i valori inalienabili del dialogo e della legalità. Gli stessi valori che Massimo D'Antona, animato da una forte passione civile, lascia a noi come eredità preziosa.

ha barbaramente ucciso il professor Massimo D'Antona. Un assassinio che ha colpito un uomo, uno studioso raffinato, le istituzioni politiche, il sindacato. Un omicidio a scopo dimostrativo, con l'obiettivo di minare alle fondamenta l'indispensabile rapporto tra intellettuali e politica, per minare un progetto di modernizzazione dello Stato e del Welfare. È stato un assassinio carico di messaggi contro tutto ciò che il professor D'Antona rappresentava. Il 20 maggio è anche l'anniversario dello Statuto dei lavoratori, una conquista di civiltà che segnò profondamente l'assetto dei rapporti sindacali e politici del nostro Paese, e Massimo D'Antona si formò in quella stagione. Nel 1980 vinse la cattedra di diritto del lavoro, come è stato ricordato, con l'opera «La reintegrazione nel posto di lavoro», ancora oggi modello di ricerca e di analisi per i giuristi che hanno a cuore l'effettività degli interventi legislativi in materia di lavoro. Nelle università di Catania, di Napoli e di Roma è stato da tutti stimato ed apprezzato per il rigore del suo metodo e la problematica profondità del suo insegnamento. Il suo lavoro scientifico è noto non solo agli studiosi, ai lettori e agli operatori del diritto sindacale, ma anche a quelli del diritto amministrativo, avendo egli contribuito, in maniera determinante, al processo di privatizzazione del pubblico impiego. Da tecnico prestato alla politica, si misurò con temi complessi, dalla riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione alla regolamentazione dei conflitti sindacali nei servizi pubblici, alla unificazione delle regole tra lavoro pubblico e lavoro privato, alla creazione di una nuova dirigenza pubblica, alla disciplina della rappresentanza sindacale nel settore pubblico. Su ciascuno di questi temi, l'impegno di D'Antona è stato quello di un intellettuale che si riconosce nei processi di riforma orientati alla modernizzazione del Paese, ed infatti la privatizzazione piena del pubblico impiego resta la sua realizzazione più compiuta sul versante normativo. L'idea di fondo era che l'effettività delle situazioni sostanziali riconosciute ai lavoratori non potesse prescindere dal confronto con le norme costituzionali, troppo a lungo neglette, che imponevano di costruire una solida coerenza tra i costi dello Stato sociale e le dinamiche della spesa pubblica. La specificità del lavoro pubblico è infatti legata al confronto non con il profitto del datore di lavoro, ma con l'interesse pubblico all'efficienza della pubblica amministrazione. E su questo binomio corre il filo della privatizzazione del pubblico impiego. L'elaborazione del Testo unico sul lavoro pubblico, il decentramento delle funzioni statali a Regioni ed enti locali e la riforma dell'amministrazione dello Stato centrale erano punti salienti della sua attività scientifica. Il più recente impegno di D'Antona è stato per il patto sociale e il piano dell'occupazione, dove pure è riuscito a introdurre la nuova cultura dell'unità delle regole tra pubblico e privato, con il Ministero del lavoro ricondotto a quel ruolo di amministrazione delle politiche del lavoro, da tempo ormai smarrito. Cari colleghi, vi sarebbero tante, troppe cose da dire su quest'uomo e su ciò che ha fatto per il nostro Paese. Ed insieme a lui è impossibile non ricordare Marco Biagi, perché uniti nella difesa dell'occupazione e legati, in maniera imprescindibile, alla creazione di uno Stato moderno e competitivo, agile nei rapporti con il lavoratore. Sono essi i martiri della democrazia, uccisi perché lavoravano per la coesione sociale e non per il conflitto di classe, uccisi perché moderni, perché sperimentavano nuove e diverse forme di partecipazione dei lavoratori al sistema produttivo italiano. Massimo D'Antona va ricordato come uomo, come studioso mite, ma profondamente determinato, come anticipatore di idee, progetti ed iniziative destinate a restare e a dare frutto. Va ricordato per non commettere nuovamente l'errore della sottovalutazione politica e culturale del terrorismo politico. Va ricordato perché, come saggiamente dice il nostro Presidente della Repubblica, deve essere scongiurato ogni rischio di rimozione e vanno riaffermati sempre i valori del dialogo e della legalità. Va ricordato per unirci alla sua famiglia, alla nostra collega ed amica Olga D'Antona, in un abbraccio forte, che faccia sentire sempre a proprio agio i familiari delle vittime del terrorismo, perché fuori posto sono gli altri, sono gli assassini, i brigatisti, i terroristi, e non loro. Lo ricordiamo, Massimo D'Antona, con profonda stima, per la tenacia e la convinzione che lo contraddistinguevano, affinché la violenza che l'ha colpito non abbia il sopravvento sui valori che di lui e con lui condividiamo. Presidente, onorevoli colleghi, incaricato dal Gruppo di parlare su un argomento che sarebbe toccato alla collega Carlino per competenza di Commissione, ho cercato una documentazione su una figura che, lo confesso, non conoscevo a sufficienza. Mi sono rivolto pertanto ad un libro, che ho qui, che ho trovato nella Biblioteca del Senato, scritto da due colleghi,

Dal libro ho ricavato la descrizione del carattere di una persona che duole davvero sapere assassinata. La nostra collega della Camera ha trovato una maniera ricca di sensibilità, intelligenza e, nello stesso tempo, estremo pudore e grande sobrietà nel delineare la figura del marito.

per affrontare uno dei problemi più difficili della società democratica. D'Antona ha affrontato da studioso e da esperto

Guardando da vicino questo argomento, si scopre che nel mondo del lavoro non c'è mai l'età dell'oro: anche quando l'economia funziona

più: fa parte della tradizione del movimento operaio e del mondo contadino, ma insieme alle parole libertà ed eguaglianza ogni tanto dovremmo ricordarla. D'Antona sapeva che nel mondo del lavoro non c'è l'età dell'oro e che, accanto alle possibilità di riscatto

Il conflitto nel mondo del lavoro non è più soltanto tra impresa e lavoratori,

D'Antona lavorava su questa materia scottante, in cui non esiste consolazione e non c'è la possibilità di

Questo tipo di materia incandescente è stato trattato da D'Antona con la prontezza dello studioso che riesce a cogliere la natura di un problema sociale ed economico e a tradurla in norma giuridica. Un mestiere difficilissimo, un mestiere che porta con sé anche il rischio della solitudine. Forse si può parlare di solitudine del riformista. Il riformista che prende una materia così bollente e cerca di trovare una via misteriosa, che non può essere il totale accordo tra le parti, perché nella democrazia il totale accordo tra le parti non c'è mai,

Credo che oggi, a dieci anni dal suo assassinio, sarebbe giusto provare a immaginare che cosa D'Antona proverebbe di fronte allo sviluppo di una realtà che lui aveva soltanto visto all'inizio: il lavoro interinale, il lavoro flessibile, il lavoro precario, oggi anche il lavoro non pagato. Proprio perché rispetto enormemente la figura di D'Antona sono costretto a ricordare, con la massima celerità, che nella trasformazione dell'università che abbiamo sotto gli occhi si immagina la copertura di più di metà dei corsi universitari, che trasmettono conoscenza e amore per la ricerca scientifica, sulla base di contratti a titolo gratuito. La domanda è molto semplice: che cosa si contratta in un contratto a titolo gratuito? Credo che uno studioso attento al sociale come D'Antona avrebbe vissuto questo vissuto questo interrogativo con angoscia crescente. Né possiamo dimenticarci che il tasso di occupazione femminile, che pure era stato fissato a Lisbona

Termino con una nota che spero non suoni stridente, ma che ci dovrebbe costringere ad interrogarci sulla nostra stessa natura: in Parlamento, su 516 coadiutori del lavoro parlamentare,

Penso che, al di là della commozione per il ricordo di una persona di straordinaria validità, noi onoreremmo nel modo migliore la memoria di Massimo D'Antona risolvendo e cancellando questa distinzione: nel Parlamento non può esserci lavoro Signor Presidente, il ricordo del professor D'Antona richiama il buio ritorno del terrorismo. Ricordare oggi la figura di quell'uomo del diritto è di estrema attualità, se solo si pensa alla pericolosa intolleranza manifestatasi a Torino quale ha fatto le spese il segretario generale della FIOM Rinaldini. Non cerchiamo strumentali analogie, cogliamo questo momento per richiamare le forze democratiche al loro ruolo di presidio della libertà di opinione, del valore forte della dialettica e della contrapposizione, ma nel contemporaneo rifiuto di ogni forma di violenza. D'Antona come Marco Biagi, accomunati nel tragico epilogo della loro vita, mettevano i loro studi, la loro scienza e la loro sensibilità al servizio dei lavoratori e sono stati vittime di sedicenti rivoluzionari che agivano per sovvertire il sistema e si spacciavano per paladini dei deboli. La lezione di D'Antona non può esaurirsi in una commemorazione ma deve essere una spia per le coscienze del Paese, per la politica, che non può tollerare agguati come quelli che furono consumati contro D'Antona e Biagi, una politica che deve evitare sul nascere le derive antidemocratiche

sempre più vicina, come lo è sempre stata, ai lavoratori, specie in questo momento delicatissimo, rivolge il suo pensiero al professor D'Antona, alla sua famiglia, ai suoi allievi che ne continuano l'opera e la cultura giuridica.

onorevoli colleghi, nel rendere omaggio alla figura di Massimo D'Antona a dieci anni dal suo brutale assassinio, prima ancora che ricordarne le qualità culturali, professionali e politiche, non posso non iniziare il mio intervento senza ricordarne le straordinarie qualità umane. La capacità di ascolto dell'altro era la caratteristica umana che più delle altre mi colpì in Massimo D'Antona. Non si trattava semplicemente di un tratto caratteriale legato alla sua educazione, che pure era presente, ma era in realtà un orientamento culturale, la volontà, ricercata costantemente e tenacemente, di portare a sintesi un pensiero unitario, una ricerca che poggiava sulla consapevolezza della complessità dei problemi connessi al passaggio epocale di fase che investiva il mondo del lavoro in quegli anni e che lo investe ancora oggi. Su questi dati di umanità, di passione politica e di cultura era basata la sua particolare capacità operativa, l'attitudine a trovare sintesi accettabili per posizioni diverse e a trasferirle rapidamente in norme giuridiche. D'Antona aveva da sempre maturato una scelta di campo, quella di stare dalla parte dei lavoratori. Una scelta per lui naturale e serena, una scelta di campo chiara che, unita alla sua capacità di ascolto, contribuì a farlo considerare interlocutore affidabile per tutti, Governo, sindacati e datori di lavoro; una scelta di campo, non di parte, che non toglieva nulla al suo spirito critico ed alla ricerca creativa di sintesi nuove al sistema storicamente definito delle tutele del lavoro. Un impegno teso alla ricerca di una nuova solidarietà ed alla ricomposizione delle frammentazioni prodotte nel campo sociale dai cambiamenti impetuosi della società e del sistema produttivo in quegli anni, nella convinzione, diceva, che «in nessuna parte del mondo il modello storico del diritto del lavoro, quale si è venuto strutturando nel corso del XX secolo, regge così com'è». D'Antona spese molti anni della sua vita - penso agli anni '90 - nella riscrittura delle regole del lavoro pubblico; anni complessi nei quali si avvertiva l'esigenza di coniugare il risanamento finanziario ad una prospettiva di valorizzazione delle risorse umane presenti nella pubblica amministrazione, verso un processo di tipo federale. È stato un lavoro lungo e complesso, che attraversò il Governo Ciampi e che fu proseguito dal ministro Bassanini nel I Governo Prodi, e di cui Massimo fu protagonista a tutti gli effetti. Un impegno che portò, dopo la stagione di Tangentopoli, a limitare il ruolo della politica nella gestione del servizio pubblico e alla privatizzazione del rapporto di lavoro. D'Antona fu protagonista e artefice della scrittura delle nuove regole della rappresentanza nel lavoro pubblico che furono determinate dall'incontro delle migliori culture riformatrici del movimento sindacale italiano; regole che ancora oggi sono alla base delle relazioni nella pubblica amministrazione, che hanno consentito la tenuta unitaria del movimento sindacale e che sono alla base degli accordi unitari per la loro estensione nel lavoro privato. Il tema della democrazia e della rappresentanza furono il «filo rosso» del lavoro di Massimo D'Antona. Era convinto, infatti, che l'unità sindacale rappresentasse un valore irrinunciabile per il movimento dei lavoratori e che tale unità dovesse poggiare su basi certe di democrazia e rappresentatività, tanto è vero che gli ultimi mesi della sua vita furono dedicati all'elaborazione di regole condivise per l'intero mondo del lavoro, a partire dal settore dei trasporti con il patto del 23 dicembre 1998. Democrazia e rappresentanza non interrogano solamente il movimento sindacale, ma la stessa politica, come ebbe modo di dire Massimo: «la domanda di diritti del lavoratore (in quanto rappresentato) porta al costituzionalismo e ai modelli della democrazia politica». A tale riguardo, proprio gli ultimi mesi della sua vita D'Antona li impiegò nella rilettura del quarto comma dell'articolo 39 della Carta costituzionale. In tal senso aveva preparato uno scritto che portava nella sua borsa al momento dell'agguato brigatista, quella borsa che fu il suo unico strumento di difesa. D'Antona riusciva a coniugare il suo impegno accademico, istituzionale, politico e sindacale con grande capacità ed intensità, nella costante ricerca della tutela dei diritti dei lavoratori e del diritto al lavoro. Nel ricercare però la salvaguardia delle tutele acquisite, non rifuggì mai dall'esplorare campi culturali difficilmente praticati dalle stesse organizzazioni sindacali e dalla politica in generale. A dieci anni dal suo assassinio e rileggendo i suoi scritti, ho ritrovato temi di estrema attualità: la rappresentanza, la difesa del diritto di sciopero e dei diritti degli utenti dei servizi pubblici, la codeterminazione l'estensione della contrattazione di secondo livello per territorio e filiera. Nel riprendere il lavoro di Massimo D'Antona e nell'assumerlo dobbiamo operare per tentare di dare nuovi diritti al lavoro precario, sia per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, sia per quanto attiene alla necessità di ricomporre un mondo del lavoro oggi globalizzato e frammentato. L'unificazione del mondo del lavoro e l'estensione della contrattazione di secondo livello erano i filoni di ricerca che Bruno Trentin investigò costringendo la CGIL ad interrogarsi, attraverso un'elaborazione nata nella Consulta giuridica di cui Massimo era l'animatore. A causa della sua caparbia e costante ricerca di politiche riformatrici, Massimo D'Antona fu ucciso dalla follia terrorista, intersecando quel filone di sangue che vide cadere prima di lui Vittorio Bachelet, Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli e, in seguito, Marco Biagi. L'ultimo ricordo che ho di Massimo D'Antona è quello di un incontro mancato. Quella mattina del 20 maggio D'Antona avrebbe dovuto partecipare ad un convegno organizzato dalla CGIL, che aveva al centro della discussione temi ancora oggi di particolare attualità: l'incentivazione alla contrattazione di secondo livello, la salvaguardia del contratto nazionale, la capacità di assumere il territorio ed il distretto quali luoghi di sviluppo e di redistribuzione della ricchezza, la democrazia e la rappresentanza sindacale. Quella discussione fu stroncata dai terroristi: quelle domande e quei tentativi di risposta sono ancora attuali. A Olga e Valentina va il nostro abbraccio.

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo molto bello che, per uno strano ghirigoro del destino,

si sarebbe dovuto svolgere. Quella mattina fu Enrico Ceccotti, un dirigente della CGIL che collaborava con Massimo nel Gabinetto di Antonio Bassolino, a chiamarmi, inorridito e commosso, per dirmi che l'incontro che stavamo organizzando con Massimo non si sarebbe potuto più tenere perché di nuovo, dopo undici anni, la sigla immonda delle Brigate rosse era tornata a colpire.

a concludersi. È bello che nel nome di Massimo D'Antona, solo qualche giorno dopo il suo assassinio, le parti trovarono la forza nobile per addivenire ad un'intesa e per dare un periodo di nuova propulsione al Paese e al suo settore produttivo più intenso. il senatore Nerozzi quando ricorda che proprio negli ultimi giorni abbiamo condiviso questa riflessione preparando i nostri ragionamenti in Commissione sui temi che adesso ci stanno occupando:

gli scritti di Massimo D'Antona, le pagine insieme dense e terse che Massimo D'Antona dedicò a quei temi e che sono ancora attualissime e ci servono da guida, da suggestione e indicazione. Come ha detto molto bene e teneramente sua moglie Olga, ieri, la ferocia oscenamente livida delle Brigate rosse non colpisce a caso, colpì un uomo che stava svolgendo un compito straordinariamente prezioso: nell'orizzonte del riformismo della sinistra italiana stava trovando una soluzione tanto più difficile quanto più esemplare per coniugare la tradizione della sinistra italiana con l'orizzonte della modernizzazione. Ci stava riuscendo e il fatto che quelle lorde mani assassine lo abbiano sottratto a questo destino ha fatto del male al Paese e al suo sviluppo civile, rattrappendo delle potenzialità che invece si sarebbero potute compiutamente squadernare e dispiegare. Mi piace ricordare di Massimo D'Antona quel tratto risorgimentale: in un Paese che troppo spesso indulge a vocazioni dannunziane, la sua vocazione era in qualche misura carducciana. Era una persona che nella compiutezza della tradizione italiana sapeva trarre condotte di grande sobrietà, schive, tenaci e determinate, ma ispirate da un senso altissimo dello Stato e del servizio a favore dello Stato come momento di condensazione dei cittadini tutti. Una tradizione che è bello ricordare oggi perché deve fungere da esempio civile per tutti e per quei giovani che ancora frequentano le nostre università e leggono le sue opere, spero traendo il tratto di un esempio che non deve essere abbandonato in nome di quegli sconclusionati malati che tante volte vogliono prevalere. Grazie Paolo, grazie colleghi, e grazie a Massimo: un uomo che è stato un onore conoscere e che è stato un dramma perdere. *(Vivi

("Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile") una serie di emendamenti «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 4 a 8 del disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.5, 4.9, 4.64, 4.0.2, 4.0.6 (limitatamente al comma 3), 4.304, 4.317, 4.318 , 4.323, 4.23, 4.313, 6.1, 6.4, 6.7, 6.46, 6.47, 6.56, 6.57, 6.630, 6.67, 6.73 (relativamente al quarto e quinto periodo), 6.310, 6.311, 6.0.5, 6.0.300, 6.0.301, 6.0.301, 6.322, 7.2, 7.7, 8.6, 8.28, 8.0.550 e 8.302. In ordine alle proposte 4.721 e 4.800a il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della copertura a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 12, In ordine alla proposta 5.22 il parere è non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che la parola "istituito" sia sostituita dalla seguente: "allocato". In ordine all'emendamento 8.704 il parere è non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della copertura finanziaria. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti dall'articolo 4 all'articolo 8, ad eccezione che sulla proposta 7.330 nonché sugli emendamenti contenuti nell'Annesso n. l».

naturalmente, e oggi è particolarmente significativa perché dalla mattinata si susseguono voci circa la volontà del Governo di porre il voto di fiducia sul decreto-legge Voglio dire, con grande franchezza, che troveremmo molto grave il ricorso al voto di fiducia; non ne vediamo in nessun modo i presupposti, e siamo fortemente tentati dal pensare che un voto di fiducia sarebbe piuttosto un *commodus discessus* perché non ci si intrattenesse in quest'Aula, con i rischi che sono collegati a votazioni dall'esito che potrebbe essere incerto, su alcune questioni essenziali, che sono alcune delle questioni che noi abbiamo, sin dall'inizio, posto con molta forza: il modello di governo della ricostruzione, una copertura finanziaria che suscita ancora perplessità e che legittima prudenza, il ruolo degli enti locali. Si tratta, tra l'altro, di un decreto del 28 aprile, che quindi scade il 28 giugno. Questo renderebbe ancora più grave il fatto che si sottraesse al Senato - e forse, di conseguenza, anche alla Camera dei deputati - la possibilità di un esame compiuto del testo. È un testo che riguarda il terremoto in Abruzzo, riguarda il Paese, riguarda ciascuno di noi, noi tutti in quanto responsabili di fronte a quelle popolazioni e rispetto a quei governi locali.

io voglio compiere un atto di piena disponibilità. Restano ancora circa 450 emendamenti; appartengono a questa parte politica soltanto 300 emendamenti che noi abbattiamo coprendo le dieci questioni che ci paiono essenziali, sulle quali ci siamo già intrattenuti e che non enumero per brevità del mio intervento, e li riduciamo a 42. Se la volontà di presentare la volontà di presentare emendamenti da parte del Governo si poggia sul numero degli emendamenti, ci aspettiamo che da parte della maggioranza, che ha presentato 150 emendamenti, ci sia un'uguale disponibilità. Signor Presidente, del tutto inammissibile e molto strano che, a fronte di questa nostra offerta (un'offerta - si badi bene - rivolta alla possibilità di avere una discussione più proficua e un miglior testo destinato alle popolazioni abruzzesi: non è un modo per piantare bandierine, altrimenti avremmo potuto praticare altre strade tra quelle che la prassi parlamentare ci offre), non seguisse il ritiro parlamentare ci offre), non seguisse il ritiro degli emendamenti da parte della maggioranza (ove possibile e ove la maggioranza lo ritenesse) e soprattutto non si rinunciasse alla pretesa del voto di fiducia.

sulla base della preoccupazione che sta emergendo nelle ultime ore in Aula per l'ipotesi di una richiesta del voto di fiducia da parte del Governo,

soltanto alcune unità per consentire l'esaurimento della discussione nella serata di oggi e concludere la votazione finale - com'era l'intesa iniziale da parte di tutti i Capigruppo - nella mattinata di domani.

- hanno manifestato l'esigenza di segnalare solo poche questioni ritenute utili ad arricchire questo provvedimento che è nell'interesse generale degli abruzzesi e non di questa o di quella parte politica. Pertanto, a fronte di questa disponibilità preventiva

la Presidenza non può che prendere atto della proposta, condivisa dall'intera opposizione, di ridurre drasticamente il numero degli emendamenti e della richiesta di sospensione della seduta, alla quale ovviamente non si sottrae.

il ritiro di tutti i nostri emendamenti.

D'altro lato, mi è pervenuta una segnalazione da parte del Governo, che ha preannunciato l'innesto di piccoli emendamenti, che sono in sede di formulazione e naturalmente non hanno carattere strategico o sostanziale rispetto

soltanto per chiederle, stante l'annuncio di emendamenti da parte del Governo, di prevedere un termine brevissimo, magari di mezz'ora,

la produzione da parte del Governo di una nuova relazione tecnica sull'articolo 14 del decreto-legge, con espresso riferimento a due emendamenti della Commissione: Questo adempimento è assolutamente necessario per pervenire ad una conclusione positiva dei lavori cosa che tutti auspichiamo.

Circa 20 giorni fa la Commissione di vigilanza Rai ha emanato un regolamento che, all'articolo 9, così suona: «Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza sulle reti nazionali, in orario di buon ascolto, le tribune politiche-elettorali

Vorrei pertanto invitarvi a una riflessione. Le donne, anche in testa di lista, forti dirigenti e forti parlamentari uscenti, sono spesso ricche solo del loro lavoro, della loro fatica e delle loro idee. Se anche il servizio pubblico, che pure attribuisce a se stesso una funzione di organizzazione funzionale alla norma di parità, a metà corso scopre di avere garantito soltanto un settimo di presenza femminile nelle tribune elettorali per le elezioni europee, allora c'è qualcosa che non funziona: la norma è vaga, è soltanto una forma di

debbano farsi carico di garantire che in questa tremenda campagna elettorale, dove varranno i blocchi organizzati e i soldi, almeno la televisione pubblica dia alle donne candidate uno strumento di pari opportunità!

una cosa del genere per visite di delegazioni straniere. Per quale motivo è accaduto ciò? Se noi, quando invitiamo delle delegazioni cinesi, adottiamo anche i loro sistemi di sicurezza, sarebbe bene che ne venissimo informati come senatori

Grazie